Comunico che in data 1[o] aprile 2021, sono stati presentati i seguenti disegni di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri della salute; della giustizia: della pubblica amministrazione; e del lavoro e delle politi- che sociali «Conversione in legge del decreto-legge 1[o] aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» (2167). dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri delle infra- strutture e della mobilità sostenibili; e della cultura «Conversione in legge del decreto-legge 1[o] aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia» Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 1[o] aprile 2021 Gentile Presidente, informo la Signoria Vostra che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero sig.ra Marina SERENI. Inoltre il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la senatrice Caterina BINI. F.to Mario Draghi».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

La seduta è tolta